nonché su quella relativa alla conciliazione tra famiglia e lavoro. In proposito è opportuno precisare che il Governo - consapevole del divario di opportunità, ancora oggi, sussistente tra i generi - ha promosso, in questi ultimi anni, specifici interventi volti ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In particolare, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009) ha messo a regime - a far data dal gennaio 2009 - la detrazione IRPEF, pari al 19 per cento, delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza agli asili nido statali, comunali o privati, su un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio iscritto. In aggiunta alle risorse stanziate, per il triennio 2007-2009, con il Piano straordinario per lo sviluppo della rete integrata dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (per un importo totale di 727 milioni di euro), il Governo ha destinato, per l'anno 2010, 100 milioni di euro in favore delle Regioni al fine di implementare, in via prioritaria, lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia nonché per la realizzazione di altri interventi a favore della famiglia. Nel corso dell'ultimo triennio inoltre è stata attivata la sperimentazione delle cosiddette sezioni primavera - sezioni nido aggregate alla scuola dell'infanzia - finanziate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Informo al riguardo che, per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, nonché per il corrente anno scolastico, il contributo dell'amministrazione che rappresento è stato pari a 1.400.000 euro.

un meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali. Il Quadro strategico nazionale ha in particolare individuato per le Regioni del Mezzogiorno quattro obiettivi, tra i quali l'aumento dei servizi socio-sanitari in favore di bambini ed anziani al fine di agevolare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. In linea con tale obiettivo, ha preso avvio nel gennaio 2009 il progetto Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio-Servizi per l'infanzia gestito dall'amministrazione che rappresento congiuntamente al Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - per il quale sono stati assegnati, per il periodo 2007-2013, 2 milioni di euro.

di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e dei servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia, l'istituzione dei cosiddetti asili domiciliari, che si avvalgono di persone adeguatamente formate che offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio. Nella medesima direzione si collocano il Piano recante il sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il Piano d'azione per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro (il cosiddetto Piano donne Italia 2020). Il primo, in particolare, ha investito 40 milioni di euro del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in finanziamenti per il telelavoro e per la formazione volta a sostenere il rientro nel lavoro dopo un periodo di congedo per maternità. Il Piano donne Italia 2020, sottoscritto dai ministri Sacconi e Carfagna, prevede 40 milioni di euro per favorire l'occupazione femminile attraverso la diffusione dei nidi familiari, il potenziamento dei servizi di cura, la creazione di albi di badanti e di *baby-sitter* appositamente formate, il sostegno economico a chi lavora da casa tramite telelavoro e gli sgravi fiscali sul lavoro delle donne del Mezzogiorno. Faccio inoltre presente che l'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010 (intitolato «Contratto di produttività»), convertito dalla legge n. 122 del 2010, ha potenziato ed ampliato - attraverso la esplicita previsione degli accordi territoriali o aziendali di secondo livello - il ruolo della contrattazione collettiva che, come affermato dall'accordo quadro del 22 gennaio 2009, costituisce il terreno fertile

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un avviso comune sulle misure a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, con l'obiettivo primario di sostenere la crescita dell'occupazione femminile. Nell'intesa si sottolinea, in particolare, l'importanza di una modulazione flessibile dei tempi di lavoro tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, nella consapevolezza che la migliore conciliazione tra esigenze produttive e quelle delle persone possa essere realizzata anche attraverso il ricorso alla contrattazione collettiva di secondo livello. Nel medesimo contesto, inoltre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali si sono impegnati a valorizzare - compatibilmente con le esigenze organizzative, produttive e le dimensioni aziendali - le buone pratiche di flessibilità e di conciliazione esistenti, provvedendo a tal fine ad attivare un tavolo tecnico per la verifica delle buoni prassi nonché delle relative azioni di monitoraggio effettuate dalla cabina di pilotaggio istituita nell'ambito del Piano Italia 2020. Nell'ambito delle misure volte a favorire la conciliazione tra famiglia e lavoro, assume altresì particolare rilievo il Regolamento adottato - ai sensi dell'articolo 9,

in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono progetti volti a consentire particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro. Informo, in proposito, che lo scorso 20 maggio è stato pubblicato il relativo avviso di finanziamento che, per l'anno 2011, ha previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia. Con specifico riferimento a quanto rilevato nel presente atto parlamentare, tengo inoltre a precisare che,

ha previsto il differimento di 24 mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di occupazione femminile - di cui alla legge n. 247 del 2007 - al fine di consentire al Governo di procedere al riordino del quadro normativo vigente. Da ultimo, colgo l'occasione per precisare che il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183 con il quale il Governo ha esercitato la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Tale provvedimento, in particolare, reca al suo interno importanti disposizioni volte a conciliare gli impegni di lavoro con i carichi familiari.

le numerose informazioni che ha fornito. Devo dire però che non trovo soddisfacente la sua risposta, perché

degli elementi peggiori della condizione economica e sociale del nostro Paese, quello del divario di partecipazione al lavoro delle donne, di cui non sto a richiamare i dati, perché sono noti, da ultimo ricordati nella relazione annuale dell'ISTAT e nell'ultima relazione del Governatore di Bankitalia. Si tratta di un elemento, voglio ricordare, non solo di grave difetto di democrazia, ma

repertorio di misure poste in essere che in realtà fanno riferimento all'attuazione di norme previgenti, quindi non inquadrano il disegno e le politiche che l'attuale Governo mettere in campo per superare questo gravissimo divario di partecipazione. Tutti gli stanziamenti di misure che lei, Sottosegretario, ha richiamato nella prima parte della sua risposta, dalla conferma delle detrazioni IRPEF conferma delle detrazioni IRPEF per le rette degli asili al trasferimento dei fondi alle Regioni per il piano dei servizi per la prima infanzia, non sono altro che la conseguenza di norme messe in campo dal Governo precedente. In particolare, la detrazione IRPEF sulla retta dei nidi è una misura messa in campo nel 2007 dal Governo Prodi ed il trasferimento alle Regioni di risorse per l'attuazione della rete dei nidi era una delle misure previste dal Piano straordinario per gli asili nido, nido, che ha subito, dal 2008 in poi, prima un blocco e poi un sostanziale definanziamento. Le risorse che sono state trasferite sono il residuo di 1,1 miliardi di euro che rappresentava la prima quota di finanziamento messa in campo dal Governo Prodi di un piano che avrebbe dovuto essere finanziato in termini incrementali negli anni successivi e che invece è stato bloccato. Ancora, avevamo chiesto di conoscere in maniera precisa quali fossero le azioni e, soprattutto, le risorse messe in campo dal Governo a finanziamento di quello che anche lei ha qui rappresentato come il principale strumento di intervento per garantire l'aumento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, che è individuato dal Governo Berlusconi nel cosiddetto Piano

di dimensioni straordinariamente piccole in rapporto alle misure che, viceversa, a partire dalla sottoscrizione del protocollo per il *welfare* per il 2007, poi recepito in norma di legge, erano state destinate all'attuazione delle misure di conciliazione e di sviluppo.

del 2000, per il quale sono stati, con bando che lei ha ricordato, recentemente mobilizzati 15 milioni di euro, che fanno parte però della dotazione del 2007. Al riguardo, ricordo che dal 2007 non vengono erogati fondi per l'implementazione delle politiche di conciliazione delle imprese. è il rifinanziamento, per l'appunto, del Piano nazionale per gli asili nido, nonché delle misure di defiscalizzazione ad esso collegate, che ancora fanno riferimento alle misure di defiscalizzazione messe in campo con la finanziaria per il 2009. Non c'è quindi niente di nuovo, se

In proposito, è opportuno ricordare che tale materia ha subito importanti modifiche a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) che, nell'intento di omogeneizzare e razionalizzare le diverse disposizioni che ne fissavano i principi regolatori, ha previsto nuove modalità per coloro che intendessero fare ricorso all'istituto della ricongiunzione. Il complessivo sistema in tal modo delineato comporta che i lavoratori i quali non potranno raggiungere i requisiti minimi per il conseguimento della pensione nei fondi di appartenenza potranno ricorrere alla ricongiunzione, sostenendo un onere variabile a seconda della situazione previdenziale di ciascuno. Con specifico riferimento alle categorie dei lavoratori elettrici e telefonici, iscritti ai relativi fondi (soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2000), preciso che le stesse, a seguito dell'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, non possono più ricongiungere gratuitamente all'Assicurazione generale obbligatoria i periodi contributivi maturati presso il fondo di appartenenza e, una volta cessata l'iscrizione al fondo medesimo, trasferire gratuitamente la propria posizione assicurativa In particolare, per effetto delle nuove disposizioni, i soggetti cessati dal servizio, in presenza dei requisiti per il diritto a pensione, possono continuare a trasferire la contribuzione nel fondo pensioni lavoratori dipendenti ma solo a titolo oneroso. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori cessati senza diritto a pensione, occorre distinguere tra quelli cessati prima o dopo il 30 giugno 2010. Questi ultimi, infatti, per far transitare la propria posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria devono avvalersi necessariamente del trasferimento a titolo oneroso; nel caso, invece, di soggetti cessati prima del 30 giugno, si sono create situazioni diverse nei confronti dei lavoratori elettrici rispetto a quelli telefonici. In particolare, per i lavoratori telefonici interessati da una norma che consentiva la costituzione d'ufficio a titolo gratuito della contribuzione del rispettivo fondo continuano ad avvalersene purché abbiano cessato, alla data del 30 giugno 2010, l'iscrizione al fondo, telefonici senza diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Per i lavoratori elettrici cessati alla data del 30 giugno dall'iscrizione al relativo Fondo che abbiano maturato o meno i requisiti pensionistici, ma che entro la stessa data abbiano presentato la relativa domanda di costituzione della posizione assicurativa, continua ad applicarsi la normativa previgente. Ricordo altresì che - sulla base delle disposizioni normative vigenti - i soggetti in esame possono usufruire, in alternativa e in presenza dei requisiti richiesti, dell'istituto della totalizzazione. Ciò premesso - preso atto delle indubbie ripercussioni che tale riforma ha prodotto sul tessuto sociale nonché della necessità di consentire un adeguato riconoscimento previdenziale all'attività prestata dall'assicurato nell'intero arco lavorativo tengo a precisare che l'amministrazione che rappresento ha assunto l'impegno di procedere, attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, alla individuazione di nuove ipotesi di riunificazione che consentano la valorizzazione delle posizioni assicurative possedute dal lavoratore in più gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. In proposito, rendo noto che, a conclusione dei lavori del tavolo tecnico, sono state individuate alcune linee di un possibile intervento normativo, tra le quali segnalo: la creazione di un nuovo strumento di valorizzazione delle posizioni assicurative - alternativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione - finalizzato al conseguimento del trattamento di sola vecchiaia o, in alternativa, di vecchiaia e di anzianità

riunione dei periodi contributivi non coincidenti maturati in diverse gestioni previdenziali che presentino una durata inferiore ai tre anni.

chiedo di poter prendere visione in dettaglio della risposta per iscritto, poiché si tratta di materia molto complessa, e le ultime informazioni che lei ha inserito nella risposta ritengo che abbiano bisogno di un vaglio più preciso. Il problema da noi posto, lei ha richiamato all'inizio, descrivendo la situazione creatasi, è in qualche modo, se non ho male inteso, preso in carico dalla istituzione di questo tavolo tecnico, a cui, però, chiediamo venga dato rapidamente seguito. Sappiamo che sono allo studio ipotesi che lavorino sul tema della ricongiunzione di tutte le posizioni

il raggiungimento e il ristabilimento di un punto di equità che era stato violato in maniera gravissima dal decreto n. 78 del 2010. Lei ha richiamato in maniera la proposta o, meglio, l'obbligo, che quella norma contiene, alla ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi. Ore oltre alla ingiustizia generata dalla necessità di versare risorse ulteriori per rimettere insieme il proprio percorso di carriera - e, lo voglio sottolineare, non solo per acquisire le migliori condizioni di trattamento pensionistico (che, comunque, sarebbe obiettivo largamente condivisibile condivisibile e accettabile), ma semplicemente per raggiungere, il più delle volte, i requisiti minimi per il pensionamento - si è generata, a tutt'oggi, una situazione di iniquità inaccettabile, sia per l'entità e l'ammontare dei versamenti integrativi, resi necessari dalle ricongiunzioni, sia perché per molti lavoratori la nuova normativa non consente il raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Quindi avrebbe costretto, e costringerà, se non diversamente modificata, molte persone a rinunciare a una quota della propria carriera contributiva. In alcuni casi si hanno perdite di contributi che arrivano a 20 anni, per via dei vincoli imposti alla ricongiunzione di tutti i periodi. Sottolineo che in molti casi la parcellizzazione di queste carriere di queste carriere è stato indotto non già da scelte personali, ma dalle vicende che hanno interessato le ex aziende di Stato poi privatizzate e spezzettate. Tali lavoratori, quindi, subiscono una penalizzazione gravissima, che andrà a detrimento del loro trattamento

Auspico, signor Sottosegretario, che il tavolo tecnico non si limiti a repertoriare i casi in essere, ma assuma posizioni, che peraltro si sono già manifestate in sede parlamentare e che hanno trovato condivisione trasversale, che vadano nella direzione della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi della carriera lavorativa di ciascuno, senza alcun onere, presso un'unica cassa, secondo il principio che nessun contributo, per nessuna giornata di lavoro, deve essere perso, perché a tutti gli